l'anniversario della scomparsa del senatore Giuseppe Maggiore, che si è spento il 2 marzo 2010 a causa di un brutto ed improvviso male che lo ha sottratto ai suoi cari e a tutti noi. Molti di noi hanno conosciuto di persona il senatore Maggiore che si è sempre distinto in questa Assemblea per il tratto signorile oltre che per la rettitudine, lo spirito di collaborazione e soprattutto - e vorrei sottolinearlo - un altissimo senso dello Stato e delle istituzioni. Nato a Lipari, in Sicilia, nel 1930, egli ha speso la vita al servizio del Paese, culminando la carriera come prefetto di Verona dal 1988 al 1995 e, prima ancora, come prefetto di Vicenza e di Rovigo. Eletto senatore a Verona nella XIII legislatura, a Palazzo Madama ha ricoperto l'incarico di Segretario della Commissione affari costituzionali e poi della Commissione affari esteri, nonché di membro della Commissione speciale per l'infanzia e della Commissione consultiva per la riforma della pubblica amministrazione. Molti di noi ricordano l'impegno e il contributo del senatore Maggiore in Senato, che furono sempre coerenti con la sua devozione di servitore dello Stato. A Verona, come testimoniano numerosi colleghi, ha lasciato un ricordo indelebile per la costanza, l'amore e l'efficacia con cui per tanti anni ha contribuito al bene della città. Vorrei quindi cogliere l'occasione per rivolgere un saluto affettuoso alla consorte Rosanna e ai figli Daniele e Antonino e ricordare ancora una volta con molta stima e considerazione il senatore Maggiore.

viene presentato per la prima volta al Parlamento quale primo atto del semestre europeo, cioè del nuovo ciclo di finanza pubblica concordato in sede europea: uno spazio al tempo stesso fisico e temporale dove iniziare a organizzare, all'interno di un unico processo politico, indirizzi ed impegni comuni e coordinati. Con l'approvazione del Patto per l'euro da parte del Consiglio europeo alla fine del marzo 2011, gli Stati dell'Unione europea hanno fatto un passo in avanti verso la creazione di un sistema di politiche fiscali integrate e coordinate. L'Italia, primo fra i Paesi europei, si è adeguata al nuovo calendario apportando alcune modifiche alla recente riforma della legge di contabilità. Il Documento in esame rappresenta quindi il primo passo di questa nuova e complessa architettura istituzionale e si compone di tre sezioni: il Programma di stabilità, il Programma nazionale di riforma (entrambi da trasmettere all'Unione europea) e le Analisi di Finanza pubblica. Si tratta di un documento articolato e pieno di contenuti, che merita un'analisi approfondita e sistematica. Per la prima volta il Programma nazionale di riforma, che riflette gli impegni del Paese per l'attuazione degli obiettivi di Europa 2020, viene presentato insieme al Programma di stabilità, per dare una visione organica dell'interazione tra le politiche economiche e fiscali e le politiche strutturali, riflesso, questo, della convinzione che nell'interesse del Paese non esistono i presupposti per una crescita duratura ed equa senza stabilità del pubblico bilancio. Il ministro Tremonti lo ha sintetizzato efficacemente con la formula: crescita senza deficit. Questa è la sintesi del Documento che andiamo a discutere in queste giornate. Il quadro macroeconomico descritto riflette la complessità del momento che viviamo, nel quale si innesta la pesante eredità del forte rallentamento economico del 2009, ma si intravedono i primi segnali positivi per il futuro. Nel 2010 l'economia mondiale è tornata a crescere a un ritmo sostenuto e nel 2011 le previsioni relative alla crescita dell'economia e all'espansione del commercio internazionale sono state riviste al rialzo dalle principali organizzazioni internazionali. Anche la crescita del prodotto in Italia, come sottolineato dal Documento, è stata vivace nella prima parte del 2010, in linea con gli sviluppi della maggior parte dei Paesi europei:

Ricordiamo tuttavia come la nostra crescita sia tutta da economia reale, senza *deficit spending*, al contrario di quanto ad esempio è avvenuto nei due Paesi citati in precedenza. La crescita è trainata dalle esportazioni, aumentate del 9,1 per cento, riflesso di un sistema economico e produttivo che continua a farsi apprezzare all'estero.

contro un magro 34 per cento delle aziende grandi. Nel triennio 2012-2014, il quadro che emerge dal Documento presenta luci e ombre. Il PIL, la cui stima è fondata su parametri di prudenza (1,3 nel 2012, 1,5 nel 2013 e 1,6 nel 2014), vede una crescita moderata ma in aumento. Anche l'occupazione e i consumi confermano l'uscita dal tunnel della crisi. L'inflazione mostra segnali che devono essere attentamente monitorati. Passando alla finanza pubblica, la chiusura dell'anno 2010 ha evidenziato un risultato migliore dell'indebitamento netto in rapporto al PIL, rispetto ai risultati 2009 e anche a quanto stimato nel precedente aggiornamento di settembre. L'indebitamento netto nominale del 2010 è stato pari a meno 4,6 per cento, inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto a quello dell'anno precedente. La pressione fiscale ha registrato una riduzione pari al 42,6 per cento, inferiore quindi di cinque decimi di punto rispetto al 2009 (di questi tempi ridurre la pressione fiscale certamente non è poca cosa). L'andamento della spesa evidenzia un forte rallentamento della spesa corrente primaria e una riduzione sia della spesa per interessi che di quella in conto capitale. Quest'ultimo dato sconta anche l'elevato livello di spesa in conto capitale realizzato nel 2009 rispetto all'anno precedente. L'andamento del debito ha risentito ancora in parte della crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2008 e che ha coinvolto gravemente, in particolare nel 2010, molti Paesi europei, come la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo. Bisogna dare atto che tali risultati

Bisogna dare atto che tali risultati confermano il successo della politica di rigore sui conti pubblici perseguita dal ministro Tremonti e sostenuta dal Parlamento. I dati esposti provano che le correzioni adottate in sede legislativa sulla spesa forniscono segnali positivi e mostrano la strada da imboccare per realizzare gli obiettivi ambiziosi che questa maggioranza si pone,

obiettivo sicuramente ambizioso (ricordo ai colleghi che l'unica volta che abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio è stato con il mitico Marco Minghetti nel lontano 1876), ma necessario e ineludibile. In termini strutturali, tali obiettivi confermano un miglioramento di 0,5 punti di PIL nel 2011 e di 0,8 punti per gli anni successivi, in linea con gli orientamenti strategici per le politiche economiche approvati dal Consiglio europeo a fine marzo. Questi dati confermano l'impegno dell'Italia a rispettare il nuovo quadro di regole e di responsabilità stabilito in sede europea. Il deficit italiano scenderà sotto la soglia del 3 per cento come concordato con le istituzioni europee in seguito alla apertura della procedura per disavanzi eccessivi, mentre nel 2014 viene raggiunto un livello prossimo al pareggio di bilancio. Tali obiettivi di saldo - secondo le simulazioni presentate dai rappresentanti della Banca d'Italia - consentirebbero di rispettare la regola sul debito, qualora approvata nelle forme attualmente in discussione in sede europea. Per realizzare tali obiettivi, il Documento evidenzia che per il 2011 e il 2012 non sono necessarie azioni di correzione, in quanto i conti scontano gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010 e della legge di stabilità 2011. nel 2014 il Documento prospetta una correzione pari al 2,3 per cento di PIL cumulato. Tornerò su questo punto più avanti. Oltre al percorso di consolidamento, la finanza pubblica italiana si trova a fronteggiare ulteriori sfide ed incognite. L'impatto dell'invecchiamento della popolazione rappresenta una variabile che influenzerà sempre di più la spesa pubblica, in particolare quella pensionistica, nonché quella assistenziale e sanitaria. L'equilibrio previdenziale, ad esempio, viene messo a dura prova dall'innalzamento delle aspettative di vita e dalla ridotta natalità ormai registrata nei Paesi occidentali. Dobbiamo rispondere a tali sfide contemperando le esigenze di sostenibilità della finanza pubblica con le tutele sociali che caratterizzano i Paesi occidentali. Numerose incertezze provengono inoltre dal settore bancario e finanziario, dove la nuova regolamentazione internazionale dettata da Basilea 2 e 3, anche in seguito alla recente crisi sistemica dei mercati finanziari, richiede impegnativi piani di ristrutturazione e disponibilità di capitale che rischiano di porre sotto tensione il sistema delle imprese, già in sofferenza per le difficoltà recenti connesse con il rallentato ciclo economico,

Sui mercati finanziari pesano ancora le incognite dei debiti sovrani che, come ormai riportato su tutti i quotidiani, e non solo nelle sedi tecniche, inizia a interessare anche economie fino ad ora insospettabili. Pur nella preoccupazione del momento - grave, considerate le interrelazioni sistemiche dei mercati globalizzati - occorre tenere conto che l'Italia è rimasta al di fuori delle operazioni speculative grazie alla saggia politica di rigore sui conti pubblici e alle caratteristiche patrimoniali delle nostre famiglie e imprese, riflesso dal limitato debito del settore privato. Tornando ora alle tematiche di finanza pubblica, l'indirizzo del Governo prefigura la necessità che la correzione prevista per gli anni 2013 e 2014 sia diretta sulla spesa primaria, senza tuttavia sacrificare la spesa necessaria a favorire la crescita economica. Il Governo afferma esplicitamente che si impegna a mantenere il prelievo fiscale allo stesso livello registrato nel 2010. Tale quadro prefigura un impegno gravoso, ma necessario per consentire al Paese di realizzare finanze pubbliche sostenibili, che permettono di assicurare un futuro equo alle nuove generazioni. Sarà necessario a tal fine uno sforzo di tutti i soggetti istituzionali affinché le azioni intraprese riducano gli sprechi e le inefficienze e mirino ad aumentare il livello di produttività dell'amministrazione pubblica, sempre nell'ottica di garantire il miglior servizio al cittadino. Il federalismo, ne siamo certi, contribuirà a tali obiettivi, creando gli stimoli per un uso più efficiente delle risorse pubbliche. Questo è il motivo per cui è essenziale completare al più presto il processo di attuazione delle riforme già approvate, sia quella municipale che quella regionale, affinché gli enti territoriali possano godere di un grado di autonomia di entrata e di spesa sufficiente a finanziare tutte le funzioni loro assegnate. È inoltre indispensabile pensare a dei meccanismi di incentivo che premino le realtà territoriali più virtuose, pur considerando l'esigenza di definire un sistema di perequazione delle risorse a favore dei territori a minor capacità fiscale. Ma la vera sfida del risanamento è incentrata oggi sulla crescita. Molti punti del Documento in esame presentano una visione strategica di medio periodo sui principali temi di attualità economica. la riforma della tassazione. Nel quadro presentato dal Governo, sostenuto da tavoli di specialisti e tavoli di concertazione con le parti sociali, si prefigura il passaggio da una forma di prelievo centralizzata ad una decentralizzata, nonché l'obiettivo di puntare sul passaggio della tassazione dalle persone alle cose. Il nuovo sistema tributario deve inoltre mirare a minimizzare le distorsioni legate al prelievo al fine di aumentare l'efficienza e di ridurre gli effetti di disincentivo sull'offerta del lavoro e sull'allocazione del capitale. A tal fine, sarà necessario semplificare la complessa giungla di norme e di procedure che attualmente rende il nostro sistema fiscale tra i più difficili e costosi da amministrare. E' importante fornire soluzioni ai giovani per il futuro, strumenti di stimolo all'occupazione tramite la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile di lungo periodo, promuovendo la "flessicurezza", rivedendo le norme relative alla contrattazione del lavoro e e pensando ad una politica di tassazione del reddito volta a minimizzare la distorsione nell'offerta di lavoro. Importanti sono anche le azioni dirette a ridurre il lavoro sommerso. Numerosi altri temi di estremo rilievo sono presenti nel Documento, tutti finalizzati ad affrontare i nodi strutturali che caratterizzano la nostra economia. Tra questi, le politiche di istruzione e di incremento del capitale umano, attraverso il completamento della riforma della scuola e dell'università, affinché sia premiato il merito e venga rafforzato l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché la riforma della pubblica amministrazione, che deve puntare alla semplificazione del complesso apparato burocratico che ancora impedisce al cittadino di ottenere l'accesso ai propri diritti e interessi in tempi rapidi. Deve quindi essere rafforzato l'istituto del silenzio-assenso da parte della pubblica amministrazione e devono essere velocizzate le procedure per l'apertura di nuove imprese e la realizzazione di opere pubbliche e di edilizia privata. Spero ci sia il tempo, in sede di discussione e di confronto, di approfondire le numerose implicazioni di tali temi, che sulla loro soluzione si gioca il futuro del Paese. Già in Commissione abbiamo avuto modo di svolgere un dibattito molto serio ed approfondito, con contributi

quella che mi accingo a presentare sarà davvero un'integrazione della relazione scritta perché ho pensato che il tentativo di riassumere giudizi e proposte contenuti nella relazione scritta avrebbe solo peggiorato il prodotto. Pertanto, ammesso mai che vi sia qualche collega interessato a farlo, rinvio alla lettura della relazione scritta, a presentare di seguito soltanto qualche ulteriore osservazione.

nazionale di riforma, che la politica italiana, tutta, avrebbe usato questa occasione per dimostrarsi vitale, impegnandosi nella costruzione del futuro del Paese: un'occasione per la politica italiana per dimostrarsi non autoreferenziale, ripiegata a parlare di se stessa a se stessa, in un vociare inconcludente e rissoso che ha trasformato il dibattito politico italiano in una sorta di estenuante *reality*. Si poteva sperare, ma l'occasione è stata perduta, prima di tutto, a mio giudizio, per responsabilità del Governo. «Andiamo avanti», hanno detto Berlusconi e Bossi nell'autunno e nell'inverno scorsi, a conclusione della fase che sembrava portare alla crisi di Governo. Il Documento di economia e finanza e il Programma nazionale di riforma erano un'occasione unica, dunque, per dire al Paese e all'Europa - e anche magari all'opposizione, perché no - verso dove andare con quali obiettivi e attraverso quali precise scelte. Ecco invece il DEF annunciare per il 2013 ed il 2014 una manovra correttiva dei conti pubblici per 2,3 punti di prodotto, tutta dal lato della spesa, al fine di conseguire l'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio nel 2014. Entità della correzione (questa è una prima valutazione su cui si insiste molto nella relazione tecnica): nella relazione tecnica): è obiettivo che noi condividiamo. Ma quali sono, questo è il punto, le scelte da compiere subito, per fare in modo che possano conseguire effettivamente nel 2013 e nel 2014 i risultati programmati? Su questo, nel Documento di economia e finanza è buio pesto, silenzio assoluto. È il segno,

progettare e mettere in atto una manovra anticipata di correzione dei conti valida per il 2009, 2010 e 2011. Non importa, importa, ai fini del ragionamento che sto sviluppando, che la manovra fosse fatta di scelte che ovviamente noi non abbiamo condiviso e non condividevamo; rileva invece, ai fini della discussione che sto facendo, che quella manovra fosse precisa negli obiettivi, definita nelle specifiche scelte atte a conseguirli, dotata della necessaria profondità temporale, cioè riferita a un periodo di tempo medio-lungo. La forza politica di allora ha lasciato il posto all'attuale debolezza e precarietà del Governo: ecco perché il Governo, con il Documento di economia e finanza, mostra di subire passivamente i vincoli che vengono dal Patto euro plus; promette la manovra perché vi è costretto dal Patto che ha concluso in sede europea, ma non la qualifica. Il Governo arriva al punto, signor Presidente, in piena fase di attuazione del federalismo fiscale, di violare apertamente la legge di contabilità - un problema a cui, per la verità, nel corso di questa discussione, bisognerebbe

se il Documento - come nel caso specifico - prevede una manovra, in essa devono essere indicati, per il contributo che partitamente le danno, i cosiddetti sottosettori della pubblica amministrazione, cioè lo Stato centrale, il sistema delle autonomie locali, gli enti di previdenza.

nel 2011, le scelte necessarie, la riduzione della spesa corrente non si determinerà nel 2013 e 2014 e l'indebitamento strutturale ridotto allo zero, cioè l'obiettivo del pareggio di bilancio, non verrà conseguito, mettendo a rischio la stabilità del sistema Italia, la sua credibilità nel contesto europeo e globale: è un rischio che può costarci molto, perché può tradursi in un aumento dello *spread*, cioè della differenza tra i tassi d'interesse dei titoli di Stato tedeschi e i tassi d'interesse dei titoli di Stato italiani, con conseguenze devastanti per la finanza pubblica e per il nostro sistema economico. Per questo è il punto - il Governo non sceglie? Per quale motivo il Governo non decide? Dice che ci vuole una manovra, ma rinvia nel tempo la sua definizione concreta. Le polemiche che squassano la maggioranza - tra la Libia e le politiche per l'immigrazione, tra violenti critici e acritici difensori del Ministro dell'economia - forniscono una risposta persino in termini di cronaca quotidiana, di cronaca spicciola. Più a fondo però questa incertezza, questo non decidere, questo rinviare nel tempo nasce dal fatto che ormai giungono al pettine nodi essenziali, che le forze politiche del centrodestra, ma soprattutto la *leadership* del centrodestra, non riescono più a sciogliere. Per esempio - il quesito fondamentale - l'Europa del Governo Berlusconi è quella federazione basata sulla doppia componente nazionale e regionale di cui scrive - potete controllare se ho citato correttamente - il Ministro dell'economia nella premessa del Documento di economia e finanza, una posizione politica assolutamente condivisa da noi e di portata storica per il nostro Paese, oppure è quell'Europa che sto citando un altro Ministro molto importante del Governo Berlusconi - ci lascia soli e di cui - altra citazione - «tanto varrebbe fare a meno»? È il ministro Maroni che parla esattamente in questi termini. E l'immigrazione? L'immigrazione è quel fenomeno che, se ben governato e gestito con l'integrazione, l'istruzione, il durissimo contrasto senza quartiere alla clandestinità, può rendere credibili nel medio periodo gli obiettivi di crescita del prodotto e di sostenibilità del debito pubblico su cui è fondato il Documento di economia e finanza, come proprio quest'ultimo afferma, o l'immigrazione è quel *mix* di faccia feroce, intolleranza culturale, incentivo alla clandestinità e - attenzione, colleghi della Lega - garanzia di regolarizzazione, che va sotto il nome di legge Bossi-Fini? Potrei proseguire con le politiche per attrarre gli investimenti diretti esteri, che pretendono di convivere con quelle per difendere l'italianità delle imprese - vorrei sapere come fanno fanno a convivere - e con le liberalizzazioni che pretendono di sposarsi con le più tradizionali chiusure corporative e con la tutela dei monopoli, come nel settore dell'energia o, a proposito di chiusure corporative, del disegno di legge approvato dal Senato con un lavoro di due mesi sulla riforma della professione forense il cui esame, per fortuna - non so se è una scelta politica o un caso - è fermo alla Camera (speriamo sia una scelta politica, collega Garavaglia). Basteranno questi esempi per dimostrare che l'occasione del Documento di economia e finanza il Governo la perde e la fa perdere al Paese perché non ha più la forza per scegliere tra le alternative, molto radicali, di strategia che il Paese ha ormai dinanzi a sé. Lo spazio per la mediazione, per il tirare a campare, non c'è più. Bisogna scegliere, il Governo non ha la forza per farlo. Mi sbaglio? Me lo auguro. Per dimostrare che sbaglio, basterà che il Governo dica ora, in questo confronto, durante questo dibattito, quale sia la composizione e le scelte essenziali della manovra che annuncia per il 2013-2014.

Vuole durare - questo lo abbiamo capito - fino al 2013, e magari ci riesce, pure contro gli interessi del Paese, ma non vuole essere misurato su obiettivi puntuali e di lungo periodo. Che fine ha fatto la crescita al 3 per cento ogni anno rispetto all'anno precedente, di cui parlava il programma elettorale del PdL e della Lega? Che fine ha fatto, colleghi, la rivoluzione liberale di cui in quel programma si parlava?

dalla lotta all'abbandono scolastico al contrasto del rischio di povertà, dagli investimenti in ricerca e sviluppo fino al tasso di occupazione. Noi aspiriamo, secondo il Governo, ad essere i peggiori d'Europa. Non lo dico io,

per le sue capacità di cambiare il Paese? No, zero ambizioni, perché bisogna giustificare la timidezza della strategia riformatrice. E ormai gli obblighi europei questa strategia riformatrice timida la fanno emergere. Il Programma nazionale di riforma parla delle cose che si sono già fatte, e praticamente non contiene una sola indicazione impegnativa su ciò che si deve fare, ma si chiama Programma nazionale di riforma 2020, non 2011. Facciamo qualche esempio: gli ammortizzatori sociali più discriminatori d'Europa si devono usare, come dice il Programma nazionale di riforma, massicciamente in deroga proprio perché bisogna mitigarne il carattere discriminatorio. infatti, si applicano secondo la legge discriminano violentemente tra lavoratori disoccupati e lavoratori disoccupati. Questa è la realtà. Il Governo nel Programma nazionale di riforma dice che sono i migliori in Europa e che hanno funzionato benissimo. Il Programma nazionale di riforma ci promette, a proposito di ammortizzatori sociali, di conservarli tali e quali sono oggi. Le politiche per il superamento degli ostacoli alla crescita della partecipazione delle donne alle forze di lavoro sono un'altra scelta strategica. Mentre tutti nel mondo e in Europa discutono di aliquote fiscali differenziate per il reddito da lavoro delle donne, il Programma nazionale di riforma tenta di consolarci con quello che, nel gergo sportivo, si chiama «un brodino», con le quote nei consigli delle società quotate: un simbolo che prende il posto di una politica. Noi preferiamo la politica, anche se non abbiamo nulla contro il simbolo, naturalmente. Anche in questo caso, anche su questo giudizio, sull'assenza di ambizioni mi sto sbagliando? Bene, allora, la risoluzione sul Documento di economia e finanza della maggioranza ridefinisca l'insieme degli obiettivi

altrimenti, in caso contrario, si darà ragione alla tesi che sto sostenendo: zero politiche precisa e per la stabilità zero ambizioni per quanto riguarda il cambiamento del Paese nel senso della promozione di maggiore coesione sociale e di maggiore crescita. Dunque, è tutta colpa del Governo l'occasione perduta del Documento di economia e finanza e del Programma nazionale di riforma? No, non possiamo negare purtroppo, cari colleghi, che il Parlamento, opposizione compresa, ci ha messo del suo: prima, il Senato ha preso la brillante decisione di non discutere il Documento di economia e finanza nella settimana in cui doveva essere discusso e votato tramite le risoluzioni, accompagnando questa decisione con sottili disquisizioni - tipiche della politica italiana - su termini ordinatori o perentori, di per sé rivelatori del rilievo riconosciuto alle scelte politiche e programmatiche contenute, nel bene e nel male, in questi documenti. poi proseguito la Camera - che almeno la discussione l'ha fatta nella settimana giusta (diciamo le cose come stanno) e ha acquisito un merito da questo punto di vista rispetto a noi - che che ha concluso l'esame del Documento di economia e finanza con un voto che fa segnare per la maggioranza e l'opposizione un risultato numerico di decine e decine di deputati inferiore a quello registrato in tutte le votazioni dei mesi precedenti in quel ramo del Parlamento. Evidentemente, su quei temi strategici oggetto di quei voti, maggioranza e opposizione investono molto, politicamente. Sul Documento di economia e finanza e sul Programma nazionale di riforma 2020, maggioranza e opposizione investono di meno. Possiamo approfittare di un errore, il ritardo con cui svolgiamo questa discussione, per porre un parziale rimedio? Ormai non ci spero più, signor Presidente, ma provo lo stesso ad avanzare una proposta. La risoluzione della maggioranza, che su questo potrebbe essere votata anche dall'opposizione, impegni il Governo ad introdurre subito, prima dell'estate, nella legislazione nazionale, come dice il Patto euro plus, le nuove regole per la decisione e la gestione della finanza pubblica definite in sede europea. Nella relazione scritta affronto diffusamente il tema, anche con proposte tecnicamente definite. Il Governo, nel Documento, si impegna a modificare a questo proposito la Costituzione, la Costituzione, e noi non abbiamo ragione di contrastare questo intento. Ma perché, signor Presidente, rinviare a domani quello che, fatto subito, introducendo queste regole nella legge di contabilità, potrebbe migliorare il merito di credito del Paese, rendendo più più sicuro ed anche un po' meno irto il cammino verso la stabilità? Infine, un'osservazione sullo squilibrio crescente tra le conoscenze e la capacità di analisi tecnica di cui dispone - ed è un bene crescente il Governo e quelle di cui dispone il Parlamento. C'è una novità molto positiva che voglio sottolineare ai colleghi, perché forse non è stata pienamente avvertita. La capacità di analisi e di elaborazione dei dati del Governo, in particolare delle strutture del Ministero dell'economia, è molto cresciuta. È testimoniata, ad esempio, dalla qualità dei test di sensitività al diverso andamento dei tassi di interesse o dell'immigrazione cui sono sottoposte le politiche politiche di rientro dal debito o quelle di sostegno della crescita. Ad esempio, colleghi, sapevo che un forte flusso di immigrazione regolare è indispensabile, da qui alla metà di questo secolo, per un adeguato ritmo di crescita del prodotto e per la correlata sostenibilità del debito, ma, lo confesso, non avrei mai immaginato quello che c'è scritto nel Documento di economia e finanza, data anche la composizione del Governo: vale a dire che le dimensioni di questo flusso, assunte nello scenario base del Governo, dovessero essere quelle fissate nel Documento di economia e finanza, cioè 221.000 immigrati in più ogni anno di qui al 2060. Questo è lo scenario base, a proposito di immigrazione, del Documento di economia e finanza nella misurazione della sensitività.

Se non lo si vuole leggere perché si preferisce affermare il contrario - cioè che non abbiamo bisogno di immigrazione buona (non di quella clandestina) e dobbiamo regolare di conseguenza la nostra iniziativa perché si vuole strumentalizzare la paura che la cattiva immigrazione determina, naturalmente possiamo evitare di fare i conti con quel dato, scritto nel Documento di economia e finanza. Il Governo, però, ha fatto la sua parte per informarci su come stanno le cose, liberi noi - se vogliamo - di infilare la testa dentro un sacco. Ma ecco il punto: a fronte di questa mole enorme di dati e di informazioni, qual è la capacità di analisi tecnica, di rielaborazione, di valutazione tecnica in chiave critica, del Parlamento? Gli sforzi del nostro Servizio del bilancio sono grandi e, anche quando sono compiuti insieme alla Camera, danno risultati di grandissimo pregio, ma cresce, signor Presidente, cresce troppo la disparità delle forze impegnate: centinaia di economisti e di analisti, da una parte,

Contrariamente a quanto si pensa, se ne gioverebbero molto di più, rispetto alle Commissioni bilancio, le Commissioni di merito, oggi strutturalmente impossibilitate

stessa opposizione, non solo per ragioni formali, essendo la prima volta che ci troviamo a discutere del Documento di economia e finanza nel quadro di un contesto europeo vincolante,

la costituzione del cosiddetto meccanismo europeo di stabilità che avrà, a partire dal 2013, una capacità di prestito di 500 miliardi di euro (simile, anzi leggermente superiore ai 700 miliardi di dollari del meccanismo americano),

e il coordinamento delle politiche economiche dei singoli Stati dell'Europa, dall'altra, per raggiungere un'unica politica economica che sia finalmente orientata alla crescita. equilibri di bilancio ed economia reale vengono messi in stretta correlazione. Non stiamo discutendo soltanto di astratte questioni di equilibrio della finanza pubblica, ma di concreti elementi riguardanti l'economia reale.

Negli anni passati, si diceva che il centrosinistra era il paladino del rigore e che il centrodestra era il paladino della riduzione delle tasse. tasse. Oggi, stando ai fatti, le questioni si presentano in maniera completamente diversa. Ricordavano i due relatori, di maggioranza e di minoranza,

Oggi si dice finalmente che l'obiettivo di fondo del Documento di economia e finanza è la crescita senza deficit. Ebbene, sono per superare i vecchi paradigmi e affermare che tutti oggi assumiamo come tema centrale la crescita senza deficit. Potrebbe essere, addirittura, se volessimo mettere anche su questo un pizzico di enfasi, la base di un nuovo patto costituzionale, sempre che non si facciano furbizie, non ci si fermi ai proclami cui non seguono mai i fatti.

Questo significa che se é proprio la piccola e piccolissima impresa che fa le migliori performance nell'*export*, noi dobbiamo dare al nostro contesto di azione un tasso di internazionalizzazione dell'impresa molto più alto di quello che stiamo dando: altro che provvedimenti protezionistici! D'altronde, guardando ai risultati di questi anni, basta domandarsi da dove venga la domanda che sostiene e può sostenere la ripresa europea e la ripresa italiana. Questa domanda viene da Paesi molto lontani, come sappiamo, dai nuovi mercati, quelli che oggi vengono chiamati i BRICS, cioè il Brasile, la Russia, l'India, la Cina,

domanda. Voglio porre una questione: mi chiedo per quanto tempo questo Paese vitale può restare vitale se la politica non si decide, finalmente, ad affrontare le questioni vere che abbiamo di fronte? La grande sfida, se i numeri sono quelli che tutti ormai conosciamo, è su come liberare le risorse per lo sviluppo. Il Documento di economia e finanza pone al pone al centro la riforma fiscale, come uno dei cardini dell'attività. Ebbene, la riforma fiscale verrà fatta, se verrà fatta (ma non si dice come), lasciando comunque il prelievo fiscale costante. E non potrebbe che essere così, perché l'Italia è un Paese con un'alta tassazione.

Ma possiamo noi restare fermi a ragionare soltanto sui saldi di bilancio, se questa è l'entità delle operazioni che vanno fatte? Non è invece giunto il tempo per tutti, maggioranza e opposizione, di ragionare sulla ricomposizione della spesa e sulla ricomposizione delle entrate?

alla composizione della spesa, ci rendiamo conto che, se togliamo la spesa per interessi (che ovviamente è molto alta in Italia, perché abbiamo un debito enorme), se togliamo la spesa previdenziale, che comunque, come tutti affermiamo, è ormai sotto controllo, al netto di questi due grandi aggregati la spesa pubblica italiana non è per niente elevata. Anzi, qualche importante

Veniva ricordato prima dal collega Morando il tema degli ammortizzatori sociali. Vogliamo aggiungere la spesa per le famiglie italiane, che è largamente al di sotto di quelli che sarebbero i bisogni? Certamente esiste il problema di rendere più efficiente la spesa della pubblica amministrazione, e anche qui bisognerebbe incidere in maniera radicale. Certamente vi è il bisogno, appunto, di rimettere sotto efficienza questi aggregati, ma basta tutto questo, o c'è anche la necessità di interrogarsi sul livello complessivo? Veniamo al versante delle entrate, per chiudere questo intervento, e anche qui voglio restare con i piedi per terra. Ricordiamo tutti che il peso delle ritenute sul lavoro dipendente e sulle pensioni

cose. Se non entriamo più nello specifico, infatti, questo diventa un *mantra*, che non significa assolutamente niente. Bisogna piuttosto ricomporre la tassazione secondo un credibile e visibile principio di progressività, da cui non possono restare esenti

distribuzione del reddito, è questo il tema: in questi anni abbiamo assistito ad una gigantesca redistribuzione del reddito alla rovescia. Se si vogliono raggiungere obiettivi ambiziosi, occorre avere coraggio, essere innovativi, rompere ogni pigrizia culturale e affrontare scelte radicali. C'è bisogno, insomma, di grande politica, altrimenti saremo costretti a dare ragione ad un grande sociologo tedesco, Ulrich Beck, che ha detto che, dopo la crisi del 2007-2008, per i ricchi c'è stata una sorta di socialismo di Stato, vale a dire il risanamento delle banche con l'intervento pubblico, cioè con i soldi di noi contribuenti, mentre si è applicato un neoliberismo spietato agli operai e ai poveri. Io credo che il nostro compito debba essere ben altro: aprire una prospettiva nuova, di forte crescita dell'economia italiana in un contesto di piena internazionalizzazione e di una nuova e più moderna distribuzione del reddito, nel senso dell'equità e dell'efficienza. Ecco perché c'è bisogno di affrontare questa occasione: non discutiamo in astratto, ma discutiamo del futuro dell'Italia. apre una nuova finestra"). Onorevoli Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo riunitasi questa mattina ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio. Rimane confermato il calendario per la settimana corrente che prevede l'esame del Documento di economia e finanza 2011 e il seguito delle mozioni sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana e sugli stabilimenti balneari. La prossima settimana, in vista delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio, l'Assemblea non terrà seduta. Le Commissioni si convocheranno in relazione ai rispettivi programmi dei lavori, con particolare riguardo ai decreti-legge in calendario. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 17 maggio per l'esame del decreto-legge sullo svolgimento delle consultazioni referendarie per l'anno 2011, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Verranno altresì discussi, ove trasmessi dalla Camera dei deputati e conclusi dalle Commissioni, il decreto-legge concernente lo svolgimento delle assemblee societarie annuali nonché il decreto-legge recante assegni *una tantum* al personale di Forze armate e di polizia. Seguirà l'esame delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre richiesto la disponibilità del Ministro dell'interno a riferire all'Assemblea nella settimana dal 17 al 19 maggio sulle problematiche riguardanti i flussi migratori, anche in relazione all'applicazione del trattato di Schengen. Si ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 5 maggio, alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli senatori. La seduta dell'Aula inizierà pertanto alle ore 10. **Calendario dei

In ogni caso, il mio Gruppo manifesta la sua netta contrarietà al calendario dei lavori, così come è stato approvato dalla Conferenza

a chiusura di questo ramo del Parlamento. Ritengo che in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, anche se, come lei sa, vi è la tornata elettorale alla fine della prossima settimana, sarebbe stato necessario e doveroso per ognuno di noi continuare a lavorare in Parlamento e non chiuderlo per due settimane. Non ritengo che diamo al Paese una buona dignitosa immagine. Certamente non diamo una immagine di laboriosità. E' un Parlamento che decide poco, lavora meno: eppure ci sarebbe tanto da fare. Voglio ricordare che, nonostante gli arresti gli arresti della giornata di oggi, continuiamo a non discutere del disegno di legge anticorruzione, del disegno di legge sulla sicurezza, ma il

ad una consuetudine che ha sempre riguardato i lavori di Camera e Senato in occasione delle elezioni amministrative. *(Applausi dai Gruppi

prospettata in Conferenza dei Capigruppo, di un calendario *light*, che desse la parvenza di una discussione su argomenti che comunque possono essere tempestivamente trattati anche la settimana successiva a quella del voto, così come è stato concordato nella Conferenza dei Capigruppo, anche con un calendario rinforzato, perché abbiamo introdotto ulteriori due decreti-legge che verranno all'esame dell'Aula, se conclusi, recuperando quindi il tempo perduto. Per la verità - non voglio introdurre una nota polemica nei confronti dei colleghi della maggioranza - per poter recuperare il tempo perduto di decreti-legge ne dovremmo esaminare almeno una ventina. Detto questo, mi sembra obiettivamente improprio che si discuta del calendario della prossima settimana: mi sembra infatti una scelta di buon senso quella di consentire ai parlamentari di svolgere la propria attività sul territorio in occasione delle elezioni amministrative, peraltro allineandosi ad una decisione che è stata adottata

chiude per consentire ai deputati di poter svolgere la loro attività, e il Senato dove, viceversa, tutto questo non sarebbe avvenuto. Forse, il collega Belisario non ha ascoltato il mio intervento... Allora forse non l'ha compreso, ma non credo. Ritengo che non sia opportuno recuperare il ritardo, creando un disagio a chi sul territorio deve spiegare le ragioni delle proprie parti politiche. Questo lo dico anche, collega Belisario, per un'altra ragione: probabilmente, se i colleghi di maggioranza vanno sul territorio anziché stare in Aula, forse avete qualche speranza di vincere in qualche Comune in più.

a svolgere la sua informativa su fatti che credo siano importanti, cioè l'idea del preannunzio di un decreto‑legge con cui il Governo si

Chiedo quindi a lei, signor Presidente, oltre che ai colleghi e a tutti i Gruppi parlamentari, di fare in modo che quel provvedimento si possa discutere alla ripresa dopo le elezioni amministrative, possibilmente il martedì pomeriggio,

Signor Presidente, a mio avviso quando l'Aula è chiamata a votare sul calendario la cosa migliore è che venga informata di come le decisioni sono state assunte nella Conferenza dei Capigruppo. in quella sede il presidente Schifani ha presentato una proposta di calendario che prevedeva un lavoro d'Aula nelle giornate di martedì pomeriggio e mercoledì mattina della prossima settimana; la questione più rilevante era la conversione in legge di un decreto‑legge che regolamenta il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie: un provvedimento che non scade

cioè il presidente del Gruppo di maggioranza relativa del Senato, chiedendo alla Conferenza di tener conto del fatto che la prossima settimana precede un'importante e delicata consultazione nazionale, di carattere amministrativo ma che riveste anche grande importanza politica, e ha domandato per il suo Gruppo la disponibilità del tempo necessario per poter condurre la campagna elettorale.

prevedesse sedute dell'Aula - non delle Commissioni - la prossima settimana. Rilevo, visto che siamo in argomento, che ben altre carenze ha mostrato nel passato l'Aula del Senato, anche recentemente, quando la settimana prima di Pasqua non abbiamo avuto la possibilità - e in Capigruppo l'ho ricordato al presidente Gasparri - di discutere del Documento

perché è bene che tutta l'Aula ne sia a conoscenza, che ho annunciato che il Partito Democratico non voterà più il calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime settimane se non verranno messi all'ordine del giorno i provvedimenti sulla corruzione e sulla sicurezza. Credo sia arrivato il momento, dopo ormai un anno e più di attesa, che questi provvedimenti vengano portati in Aula non potendo più sussistere ragioni di alcun tipo per impedirlo.

la civiltà dei nostri rapporti parlamentari). Mentre la Capigruppo era in corso, gli uffici del Presidente del Senato hanno

in Capigruppo di decidere per i lavori dell'Assemblea della prossima settimana: il presidente Schifani proponeva cioè due giornate di lavoro. Ecco, credo che soprattutto da parte del Presidente del Senato

la discussione in tempi opportuni del Documento di economia e finanza. Lo dico perché il Gruppo Misto in tutte le sue componenti, a cominciare dal presidente Baldassarri che partecipò alla Capigruppo della settimana precedente, insieme al presidente Rutelli, che poi ha avuto modo di contestare in modo plateale quella decisione (determinando l'irritazione del Presidente del Senato), aveva richiesto che la discussione di questo documento fosse tenuta la settimana scorsa, mentre abbiamo avuto una settimana vuota. Al contrario, sarebbe stato del tutto irragionevole proseguire l'attività parlamentare nella settimana che precede le elezioni, quando è normale e doveroso invece svolgere il proprio mandato politico sul territorio. Speriamo che questa vicenda, con l'imbarazzo che ne è conseguito (e questa nota del Presidente del Senato alle agenzie di stampa ne è la dimostrazione palese) serva da insegnamento. Evitiamo ulteriori occasioni in cui le incomprensioni prevalgano sulla necessità di ragionare insieme in modo condiviso.

a tantissime interpretazioni e strumentalizzazioni. Tuttavia, il Gruppo della Lega Nord, che non si è mai tirato indietro e mai lo farà quando c'è da lavorare, sottoscrive completamente quanto

Ringrazio, inoltre, il senatore Zanda per la esegesi del mio intervento in Conferenza dei Capigruppo: confermo il contenuto esatto delle mie parole da lui riferite, che è un dato assolutamente positivo, così come è positivo che egli sia d'accordo, una volta tanto, con me. con me. Di fronte alla corretta proposta del presidente Schifani, tengo a sottolinearlo, di prospettare all'Aula un normale calendario dei lavori per la prossima settimana,

del senatore Giambrone che rappresentava il Gruppo dell'Italia dei Valori (ma poc'anzi il senatore Belisario ha sostenuto qui in Aula come Capogruppo le stesse posizioni, dunque un solo Gruppo si è opposto), e lo ribadisco in Aula, che dedicarsi ad una campagna elettorale (cosa che peraltro

Trecate impegna 11 milioni di elettori è un legittimo impegno - e non un legittimo impedimento, mi verrebbe voglia di dire - perché noi siamo qui in ragione del consenso democratico dei cittadini. Ricercare il consenso, anche se sono elezioni amministrative e non politiche, credo sia una nostra funzione primaria. Quindi, non è una vacanza, ma un impegno tra la gente, quello che io ho proposto con coscienza serena alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del Senato ha preso atto che la maggioranza dei Gruppi condivideva questa opinione, e ritengo che votarla sia una cosa utile, perché affermiamo che è giusto dedicarsi alla campagna elettorale e celebrare con il

animare il dibattito sulla Conferenza dei Capigruppo a volte anche per smentire le conclusioni assunte unanimemente o a maggioranza dalla Conferenza stessa. Pensavo fosse una prassi che non dovesse essere consolidata e, per quanto mi riguarda, poiché ho assunto una posizione in Conferenza dei Capigruppo, la confermo anche in Aula.

Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, mentre tutti gli indicatori di politica economica rappresentano un Paese ingessato, con un Governo che asseconda i *desiderata* dei banchieri, degli assicuratori, dei monopolisti fiancheggiati dai capitalisti delle bollette e dei pedaggi, che si adoperano per svuotare sistematicamente le tasche

«Italia oggi», che titola: «Il Tesoro alle manovre d'autunno. Già in settembre la correzione dei conti anticipata dal DEF». Con il quarto debito pubblico al mondo, scalzati per fortuna dalla Germania, non abbiamo più l'obiettivo di un indebitamento annuale entro il 3 per cento del PIL, ma di un pareggio annuale con manovre di 40-50 miliardi di euro, che ritengo oggettivamente difficile per un Paese che non cresce, perché mortifica la concorrenza ed il mercato, stanga i consumatori e presta grande attenzione agli interessi esclusivi delle *lobby*, dei potentati economici e dei cartelli. Qui manca però il «convitato di pietra»: mi sono sforzato di ascoltare le relazioni che sono ma non ho trovato questo «convitato di pietra», questi signori banchieri che hanno prodotto la crisi e che continuano oggi a speculare meglio e più di prima. Negli anni '80 l'economia italiana è cresciuta del 25 per cento, negli anni '90 del 16 tra il 2000 ed il 2007 è cresciuta del 7 per cento, mentre gli altri Paesi dell'area euro hanno fatto meglio di noi. Abbiamo dunque una crescita inferiore a quella degli altri Paesi non abbiamo la possibilità di correggere questo DEF. La Banca d'Italia ha calcolato che, se si ritiene di concentrare la manovra per raggiungere il pareggio di bilancio tra il 2013 ed il 2014, questa non potrà essere inferiore a 35 miliardi Tra il 2010 e il 2014, la spesa pubblica, al netto degli interessi, dovrà scendere di 5,5 punti di PIL (non sappiamo come faremo). Di questi, 3,2 punti starebbero già (secondo il Governo) nel quadro tendenziale; altri 2,3 punti deriveranno da ulteriori manovre sul 2013-2014. C'è dunque un'apparente rinuncia a procedere quest'anno ed il prossimo sulla strada delle riforme strutturali, per rimandare alle calende greche, alla prossima legislatura, l'aggiustamento dei conti, mentre sarebbe necessario, anche in base alle nuove regole di *governance* europee, dettagliare la manovra correttiva. Con un debito pubblico attestato a 1.879,9 miliardi di euro a novembre, contro i 1.790,8 miliardi di euro di gennaio con una crescita secca di 89,1 miliardi di euro (più 4,9 per cento) in soli dodici mesi, che equivale ad un gravame di 31.331 euro per ognuno dei 60 milioni di abitanti, 89.519 euro a carico di ognuna delle 21 milioni di famiglie, destinato ad aumentare ulteriormente senza correzioni di rotta, non si sa come faremo a risanare le finanze del Paese. Voglio ricordare che in un anno, dal gennaio 2010 al gennaio 2011, il debito è aumentato di 89,1 miliardi di euro, oltre tre finanziarie, al ritmo di 7,425 miliardi di euro al mese, ovverosia ovverosia 1.485 euro l'anno per ognuno dei 60 milioni di abitanti, 4.242 euro sulle famiglie. In un anno quindi, oltre ai balzelli, ai costi dei servizi, al caro bolletta, al caro bolletta, al caro RC auto, alle accise sui carburanti, alla TARSU e così via, ci troveremo con un conto da pagare di quasi 2.000 euro a famiglia, mentre non si fa nulla per restituire il drenaggio fiscale ed un potere di acquisto eroso dai quotidiani balzelli, dall'aumento delle rate dei mutui e da una protervia senza pari di un sistema bancario (che nessuno evoca, forse si si è timidi) colluso con le autorità vigilanti dei "draghi" e delle "tarantole", che inventa continue stangate mascherate sulla pelle dei correntisti e dei risparmiatori stremati dal caro-banca. È di 295 euro in Italia il costo dei conti correnti, contro i 114 euro della media europea. Al contrario, questo è un Governo che soddisfa le richieste dei signori banchieri nel milleproroghe. Il signor Ministro dell'economia completa l'opera portando al Consiglio dei lo scandaloso smantellamento della legge n. 108 del 1996, per servire al meglio le richieste dei Passera e dei Mussari, con un sostanzioso aumento dei tassi soglia antiusura. E come i più fedeli camerieri dei banchieri, non contenti di aver inserito nella finanziaria del 2001 la possibilità di far indebitare gli enti locali con gli *swap*, il cui debito - secondo dati ufficiali - ha superato 80 miliardi di euro, con un rischio di controporte di 52,2 miliardi di euro, d'intesa con la CONSOB, il Ministero dell'economia prepara una nuova bozza di regolamento sui derivati, previsto dall'articolo 62 della legge n. 112 del 2008, per eseguire letteralmente le indicazioni dell'ABI. la prima bozza del regolamento conteneva disposizioni in materia di trasparenza dei contratti, prevedendo che agli enti locali fosse data un'informativa basata sull'approccio probabilistico della CONSOB e da elaborare rispettando le metodologie. Questa informativa rappresentava in modo chiaro, breve e oggettivo se e in quale misura il derivato proposto avrebbe potuto migliorare o meno la situazione dell'ente legata ad una ben precisa passività finanziaria I banchieri tornano a brindare con i derivati fuoriborsa, strumenti negoziati fuori da piattaforme e circuiti regolamentati, che sfiorano i 500.000 miliardi di euro. Lo dice l'ISDA, l'associazione mondiale degli operatori in derivati OTC (*over the counter*), stimando che il rischio di credito di questi contratti sia pari a 2.430 miliardi di euro. Se il mercato degli *swap* è immenso e senza controllo, i derivati rappresentano un possibile rischio anche per le grandi banche europee, che non differiscono nelle pratiche dai colossi americani. Ammontano infatti a 4.000 miliardi di euro i derivati nei bilanci degli istituti europei: un valore netto pari al 20 per cento degli attivi. L'allarme *swap* da 2.500 miliardi di valore netto delle perdite potenziali è pari a tre volte il debito di Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda: è con questi derivati - ripeto - che continuano a gonfiare gli utili i signori banchieri, di cui nessuno parla in quest'Aula, e me ne rammarico. Continueremo noi dell'Italia dei Valori a fare il nostro dovere di tutela dei diritti della povera gente, degli enti locali, delle imprese stangate, strozzate. Tenuto conto che il 70 per cento dei derivati fuoriborsa tra istituzioni gode di garanzie collaterali, secondo gli addetti ai lavori, il rischio di perdita per colpa dell'insolvenza della controparte è di 1.100 miliardi di dollari, circa 750 miliardi di euro: pari alla somma del *default* di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Dopo la sostituzione del Patto di stabilità e crescita siglato a Maastricht nel 1991 con il meccanismo europeo di stabilità (MES) di imminente approvazione da parte del Consiglio europeo con interventi automatici di un fondo europeo con 500 miliardi di euro, le economie più in difficoltà saranno messe sotto amministrazione controllata dalla BCE, che a sua volta sarà commissariata nella politica monetaria da Goldman Sachs, qualora dovesse essere presieduta dal governatore Draghi. Ma di questi argomenti continuo a parlare da solo. E torniamo al punto di partenza. I debiti pubblici sono cresciuti durante la crisi sistemica per gli interventi di salvataggio delle banche e di sostegno ai mercati finanziari, con i debiti privati di banche e banchieri i quali, addossati sugli Stati, sono diventati debito pubblico. Secondo la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), il sistema bancario tedesco è esposto sulla Grecia per 65,4 miliardi, sull'Irlanda per 186,4 miliardi, sul Portogallo per 44,3 miliardi e sulla Spagna per 216,6 le banche tedesche, per le quali un *crack* finanziario dei propri debitori avrebbe effetti devastanti. Il debito pubblico tedesco è diventato il terzo del mondo appunto per aver salvato le banche, ma anche le banche italiane, al di là della polvere sotto il tappeto delle distratte autorità vigilanti, non stanno messe meglio, nonostante abbiano addossato ai correntisti ed ai risparmiatori i costi dei salvataggi a rate nei decenni precedenti.

possano affrancarsi dalla dittatura morbida di banche, banchieri e manutengoli del potere economico, che lavorano per i loro esclusivi tornaconti, quindi contro gli interessi dei cittadini risparmiatori e quelli più generali del Paese. Mi spiace constatare

Questa sottovalutazione però forse è spiegabile non solo per la considerazione che questa maggioranza ha mostrato in molte circostanze per il ruolo del Parlamento,

che si è affrontata questa scadenza, una scadenza importante, un'occasione che non osiamo definire mancata per confrontarsi con il Parlamento, con le forze produttive del Paese sulle strategie economiche, finanziarie, di sviluppo, di riforme e di crescita di cui l'Italia avrebbe bisogno. Non ci sfuggono certo i dati di contesto e la crisi economica globale. È da anni che si insiste affinché i nostri documenti di programmazione economica e finanziaria siano in linea con quelli degli altri Paesi I vincoli comunitari non sono certo una scoperta del ministro Tremonti. Ci sono da un bel po' e certo diventano più stringenti ma non possono diventare in la politica economica di un Governo. I temi di risanamento e correzione dei conti pubblici sono essenziali. La riduzione della spesa lo è, ma se non si trova il modo per cominciare ad affrontare il tema della crescita e soprattutto se non si affrontano coraggiosamente le riforme necessarie e indispensabili, difficilmente ci potrà essere una seria e ulteriore correzione del debito. È per questo che cogliamo una politica che guarda al breve, è stato detto egregiamente nella relazione del senatore Morando. Non c'è neanche un settore rispetto al quale avremmo voluto essere sfidati nel merito dell'innovazione per affrontare nodi strutturali che, se riformati, avrebbero potuto portare ad una qualificazione e riduzione della spesa e, al tempo stesso, migliorare la produttività totale dei fattori del Sistema Paese. Per quanto riguarda poi il Programma di stabilità si rivedono al ribasso le valutazioni contenute nell'analogo Documento precedente e la crescita è stimata al di sotto del 2 per cento,

Dove sono le riforme strutturali attese? La riforma fiscale? Qual è il piano di riforma vero dei gangli vitali delle pubbliche amministrazioni in Italia? Dove sono le zone a burocrazia zero, lo sfoltimento di enti e livelli istituzionali, le riorganizzazioni profonde di interi settori e comparti di questo Paese, la lotta alla corruzione, la razionalizzazione di procedimenti e funzionamenti di interi apparati pubblici?

per colmare le lacune di un'ordinaria politica economica che non c'è? Dov'è la possibilità di un rilancio competitivo di questo Paese? Noi non troviamo le misure per rafforzare la concorrenza, per aprirci ai mercati e per rafforzare i punti di forza di questo Paese. Paese. Penso, ad esempio, al capitale umano, da una parte sbandierato nel Documento come una delle risorse indispensabili per lo sviluppo e dall'altra, nello stesso Documento, visto come un settore nel quale si effettueranno tagli e si dovranno rinvenire economie.

Come fa questo Governo così poco coraggioso e così poco liberale a non vedere che stiamo consegnando una generazione di giovani a sprecare i loro talenti? nostro tasso di occupazione promette di essere il più basso d'Europa. Penso in particolare alle donne, oltre che ai giovani. L'impulso del Documento sulle riforme quindi è molto modesto e non è sufficiente a condurre la crescita verso quei parametri che potrebbero ritenersi accettabili per la ripresa.

Quello che è più grave è che, anche in prospettiva, sembra vogliate portarlo solo alla stagnazione e all'immobilismo. Questa mancanza di coraggio di ridurre davvero la spesa, di riconvertirla davvero e di puntare alla crescita e alla qualità si è manifestata anche nella vostra sordità verso le nostre proposte. Vorrei chiudere dicendo che nel Patto euro plus, che impone e chiede a tutti i Paesi di attivare delle riforme, si parla a proposito dell'occupazione di riforma del mercato del lavoro per promuovere la *flexicurity*, ridurre il lavoro sommerso e aumentare la partecipazione nel mercato del lavoro. Si parla di riforme fiscali e, soprattutto, di aumentare il lavoro per le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare.

se questo Documento di economia e finanza che il Governo ci presenta è ancora valido, in quanto i termini di riferimento assunti per i calcoli della crescita e gli altri parametri a tutto quello che dovremmo comunicare a Bruxelles parlano di un rapporto tra

a dimostrazione che i dati stessi non rappresentano quelle situazioni che vengono verificate all'interno del Documento di economia e finanza, per cui non so se è il caso di rispedirlo al mittente o mittente o se ci sarà un aggiustamento dei conti e di tutto quello che viene previsto all'interno di questo Documento. Con il nuovo DEF il Governo si assume una serie di importanti impegni con l'Europa per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica. Non possiamo certo dire altrettanto per quanto riguarda gli impegni che avrebbe dovuto assumere a sostegno della crescita e dello sviluppo del Paese. Il contenuto del Programma nazionale di riforma non ci sembra all'altezza delle necessità e delle urgenze attuali dell'Italia.

detto poc'anzi) sta spingendo sempre più il sistema paese verso il declino, proprio in una fase nella quale avremmo bisogno di far fare un balzo alla crescita del nostro Paese. Solo in questo modo, infatti, possiamo sperare di ristabilire in modo strutturale e permanente l'equilibrio della finanza pubblica. Il livello del nostro debito rimane elevatissimo. Per rispettare i parametri del nuovo Patto europeo occorrerebbe ridurlo di tre punti di PIL all'anno, una cosa quasi impossibile ai tassi di crescita previsti nel Documento. E poi, solo attraverso la crescita il Paese sarà in grado di riassorbire la disoccupazione, che sta diventando una vera e propria

Il Mezzogiorno ed il Centro-Nord, che avevano già smesso di avvicinarsi negli anni scorsi, da qualche tempo hanno ricominciato ad allontanarsi come tasso di sviluppo, condizioni socio-economiche e di vita. Un Paese, una Nazione unita, quale io considero l'Italia, non può permettere che permanga un tale dualismo territoriale al proprio interno. Tra l'altro, se il Sud continua

anche il Nord certo non ride, perché dal canto suo arranca sotto i colpi della crisi economica, ma anche come conseguenza del progressivo sgretolamento del tessuto produttivo e sociale dell'intero Paese e della mancanza di un contesto adeguato agli standarddi competitività richiesti a livello internazionale. Abbiamo bisogno di tornare a occuparci dell'economia reale. Bisogna rilanciare gli investimenti produttivi, ridurre il carico fiscale sulle imprese. Bisogna far ripartire i consumi e aiutare chi ha più bisogno a non cadere nello stato di povertà. ridurre il carico fiscale sulle famiglie e introdurre meccanismi che rendano più equa la ripartizione del carico stesso tra i cittadini. riforme fiscali globali ed epocali, si potrebbe fin da subito cominciare a introdurre modifiche e cambiamenti rilevanti al nostro sistema fiscale dove questo è urgente e praticabile. Essere più pragmatici e concreti, superando gli interessi e le rendite di pochi, per occuparci delle necessità di molti. Bisogna tornare a investire in infrastrutture, in ricerca e innovazione. E questo, si badi bene, non significa solo stanziare nuove e più ingenti risorse, ma anche spendere bene e rapidamente quelle che già sono stanziate. far girare finalmente la macchina della «legge obiettivo», di cui nessuno più parla e che è entrata ormai nel dimenticatoio, anch'essa, insieme all'economia reale, vera, di tutti i giorni. Possiamo trovare le risorse attuando finalmente una vera rivisitazione della spesa. Con coraggio, dobbiamo procedere a una vera revisione dei comparti della spesa pubblica, tagliando gli sprechi. Da alcune voci di spesa pubblica corrente possono derivare risparmi cospicui con i quali finanziare gli interventi di rilancio dell'economia. Gli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione e i contributi alla produzione a fondo perduto distribuiti a pioggia a poche imprese privilegiate sono solo due esempi.

probabilmente ci terrà ancora una volta a galla, garantendo la tenuta dei conti pubblici per i prossimi due o tre anni. Ma si tratterà pur sempre di un equilibrio precario. Anche perché, con ogni probabilità, si avranno ricadute negative sull'economia. In effetti, a fronte di una manovra che per ovvi motivi tenderà a deprimere ancora di più la crescita economica, gli interventi proposti dal Programma nazionale di riforma a noi sembrano insufficienti a dare la necessaria svolta all'economia, ad accelerare lo sviluppo e a superare il dualismo territoriale italiano. Il Programma nazionale di riforma passa in rassegna i provvedimenti già messi in campo negli anni passati e riepiloga gli effetti - ripeto, presunti - dei provvedimenti medesimi. Ne sono un esempio le misure sul lavoro, le quali sono in realtà già state attuate, come per esempio la riforma della contrattazione di cui all'accordo del 22 gennaio 2009, o i provvedimenti del collegato sul lavoro varato un anno fa. In estrema sintesi, ben poco spazio viene dedicato alle proposte di nuove riforme da mettere in campo negli anni prossimi fino a fine legislatura, cioè agli interventi programmatici. Siamo di fronte a un PNR piuttosto scarno e non rispondente alla esigenze del sistema Molte delle misure programmatiche proposte sono in realtà proposte di nuovi "piani di intervento", tutti ancora da definire e quindi lungi dall'essere realizzati. Sul federalismo, l'unica vera riforma concreta che il Governo vuole portare a termine entro la legislatura, più volte abbiamo fatto notare che si sono perse molte occasioni. E poi, nonostante diversi decreti previsti dalla legge delega abbiano già visto la luce, essi rimangono tuttora problematici nella loro attuazione, visto che a loro volta rimandano ad altri numerosi interventi normativi secondari

all'euro a 1,35 e non a 1,50, come adesso, a riconoscere un modestissimo 0,4 per cento in più di crescita alle misure contenute nell'intero PNR. Siamo lontani dalla svolta di politica economica che il Paese si aspetta. Piuttosto il Governo resta aggrappato all'illusione che il traino dell'economia mondiale possa risolvere prima o poi i nostri problemi. Ma, appunto, è solo un'illusione. Nella realtà, rischiamo di penalizzare ancor più la nostra economia. E per di più, il futuro non ci risparmierà altre manovre correttive e altri maggiori sacrifici, e il tutto per garantire quell'equilibrio dei conti pubblici che in ogni caso resterà sempre precario. PRESIDENTE. È iscritta

Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo intervento nasce dal mio grande interesse verso la politica finanziaria di questo Governo, che già da molto tempo si adopera per mantenere l'Italia all'interno di un *range* accettabile che non la spinga verso il destino di altri Paesi europei, vittime delle grandi crisi che hanno purtroppo segnato questi ultimi anni. E il mio sguardo alla politica nazionale e sovranazionale non nego che sia particolarmente attento anche al fine di osservare i frutti da raccogliere a vantaggio del Meridione d'Italia, e soprattutto della Regione da cui provengo. Questo Documento, proseguendo una linea già intrapresa da precedenti strumenti normativi, innovativi della legislazione finanziaria, nasce dalla necessità di non far più i conti solo nelle nostre tasche, ma di allineare e programmare la nostra economia riflettendo noi stessi nello specchio dell'Europa. Il coordinamento è ciò che ci deve guidare perché la politica finanziaria diventi uno strumento comune e virtuoso che possa, una volta a regime, alimentare politiche nazionali e regionali altrettanto virtuose. E per virtuose intendo sia una linearità proficua e produttiva dell'economia sia un concreto e valido interesse per la cosiddetta cosa pubblica. L'Italia non può, quindi, a mio avviso, pensare di avere valore e di crescere in tutti i sensi se non supera il noto dualismo che la contraddistingue. Ormai il termine questione meridionale è di antico conio. È stato usato in ogni periodo della nostra storia di Italia unita, a volte abusato, ma ha sempre avuto una connotazione critica in senso negativo nei riguardi delle capacità del Meridione di operare a proprio vantaggio, lavorando e producendo per il bene proprio e di quello comune. Si potrebbe dire, oggi come ieri, che Regioni ed enti locali non hanno saputo sfruttare appieno le possibilità che erano, e sono state, loro concesse, nonostante il Governo Berlusconi, se guardiamo al recente passato nonché alle azioni di riforma prospettate in questo Documento, si adoperi proprio per questo: ridurre questo odioso e pesante dualismo mettendo a disposizione del Meridione tanti strumenti di varia natura, che, adeguatamente utilizzati dai governi locali, così come dai fruitori finali, non possono non portare ad un percorso virtuoso. Non mi addentro nelle tante strategie previste: il pieno utilizzo dei fondi a disposizione, la fiscalità di vantaggio, le infrastrutture, ma mi voglio soffermare su una tematica che coinvolge ogni famiglia, che mi sta particolarmente a cuore e che seguo con grande interesse nella 10a Commissione, di cui faccio parte: dell'energia, del risparmio energetico e dell'efficienza energetica. Lo sviluppo energetico del nostro Paese è di fondamentale importanza per l'intera economia nazionale, perché è necessario ridurre la dipendenza energetica dai Paesi esteri che ancora oggi si aggira intorno all'80 Lo sviluppo, liberandoci dalla dipendenza, è risparmio. Il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi mesi, in linea con le direttive europee di definizione della strategia energetica nazionale, dal decreto sulle fonti rinnovabili al terzo pacchetto energia, porta alla definizione di una politica energetica che deve innanzitutto individuare i soggetti rilevanti: istituzioni, imprese e cittadini, e le azioni da perseguire, il quadro normativo, l'incentivazione, l'educazione e soprattutto la sensibilizzazione. In particolare, mi preme sottolineare che le Regioni del Sud Italia hanno una grande potenzialità in materia di energie rinnovabili: sole, vento e biomasse. queste Regioni rivestono un ruolo determinante nell'individuazione delle iniziative più specifiche, utilizzando le tecnologie più moderne e innovative, poter sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie rinnovabili, incidendo positivamente sull'ambiente e sull'economia nazionale. Ma, per tornare ad un discorso più generale, l'Italia ha saputo evitare di rimanere vittima delle varie crisi economiche mondiali o, almeno, è riuscita a limitare i danni grazie ad una politica di larghe vedute, fondata su una diversificazione delle azioni e ad una attenta visione delle potenzialità nazionali. Anch'io, come persone molto più qualificate in campo economico, penso che molto di questo merito sia stato e sia dovuto, alla capacità intrinseca degli italiani di risparmiare, nonché alla capacità dimostrata di mantenere più stabile possibile l'apparato produttivo, soprattutto delle piccole e medie imprese. Quindi, è proprio qui che, secondo me, dobbiamo appuntare la nostra attenzione: su questa capacità, direi, genetica, che porta il popolo italiano a sapersi adeguare al benessere, come anche alla crisi. deve essere il nostro punto di forza, e ben vengano, quindi, tutte le iniziative che favoriscono il risparmio, a partire dalla fiscalità, per arrivare alla perequazione energetica, così da mettere a disposizione di noi tutti strumenti per accantonare risorse da utilizzare nei momenti di crisi, traducendo in vantaggio personale, cioè nazionale, quell'arte di arrangiarsi che, a volte, ha fatto sorridere più di una persona. Voglio ricordare che con l'azione di questo Governo in Italia non c'è stata crisi dei mutui, né del mercato immobiliare. E le stesse banche italiane hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, quando molte banche estere chiudevano, aiutate proprio dal risparmio delle famiglie italiane. L'Italia, che prima della grande crisi aveva il più alto rapporto tra debito pubblico e PIL, non è stata colpita dalla crisi debitoria dell'eurozona. E l'azione, anzi le azioni, del nostro Governo hanno fatto sì che la lettera «I» dell'acronimo dispregiativo PIGS non fosse l'Italia, anche se naturalmente ci dispiace molto per l'Irlanda che vi è incappata. Termino qui il mio discorso, ribadendo il mio totale apprezzamento nei riguardi di una politica generosa e lungimirante che ci sta facendo aggirare molti ostacoli, e non solo in campo economico.

Intendo in primo luogo soffermarmi su quella che a mio avviso ha assunto le sembianze di una vera e propria piaga sociale: la disoccupazione, che deprime e affatica i giovani di oggi, costringendoli spesso a a lasciare il nostro Paese per recarsi in altri Stati in cui poter esercitare la propria professione. Si tratta di un fenomeno ormai largamente diffuso, che è sotto gli occhi di tutti. È un peccato, perché un Paese che non guarda ai giovani non crede al futuro. Oggi siamo chiamati ad offrire alle future generazioni le stesse condizioni di cui noi abbiamo usufruito, per restituire la speranza per il loro domani. Come ha scritto una giovane filosofa vivente,

Possiamo analizzare la politica che la maggioranza ha intenzione di intraprendere per favorire l'occupazione giovanile. La soluzione proposta è quella di puntare sui contratti di apprendistato, strumenti che, a detta del Ministro dell'economia, rappresentano il tipico e conveniente contratto di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro grazie alla semplificazione regolatoria e all'efficacia della formazione in ambiente lavorativi. Ma questo obiettivo, condivisibile, come sostengono però autorevoli economisti, da solo non risolve il dramma della precarietà ma, paradossalmente, rischia di arrecare ulteriori e gravi pregiudizi ai nostri giovani lavoratori. Non possiamo, infatti, ignorare l'uso distorto che di fatto ha assunto l'utilizzo dei contratti di apprendistato da parte delle aziende, collocando la giovane forza lavoro in una situazione di precarietà e di sfruttamento economico della propria attività professionale. Sono fatti di comune conoscenza, ed è per questo che ci attendiamo che il Governo compia un passo ulteriore per tutelare i giovani lavoratori. Per non tradire le manifeste buone intenzioni, il Governo, ad esempio, dovrebbe intervenire con una disciplina specifica e puntuale in grado di regolamentare in modo rigoroso il ricorso da parte delle aziende ai contratti di apprendistato, predisponendo un meccanismo di controllo *ex ante* ed *ex post* per verificare l'applicazione concreta di questo strumento contrattuale e soprattutto dovrebbe rivedere l'intera disciplina dei contratti atipici, che sono un'infinità e creano una sorta di delusione, di precarietà e di mancanza di futuro. Occorre, infatti, garantire un utilizzo dell'apprendistato che sia conforme alle finalità annunciate e che non si traduca in un ulteriore *escamotage* giuridico che autorizzi le aziende a sfruttare il lavoro prestato dai nostri giovani. Se non si intervenisse anche in questa direzione, si correrebbe il rischio di aggravare la posizione lavorativa dei giovani. Secondo i dati elaborati dall'OCSE, il 44,4 per cento dei giovani italiani è privo di un lavoro stabile; secondo i dati ISTAT, nel 2010,

questo dato percentuale è aumentato dello 0,3 per cento. La precarietà e l'assenza di lavoro provocano inevitabilmente un drastico e preoccupante calo delle nascite: secondo stime accreditate, i nati nel 2010 sono stati 557.000 (da cui deriva un tasso di natalità pari al 9,2 per 1.000 residenti), ben 12.200 in meno rispetto al 2009. I nostri giovani non coltivano più il sogno di fare figli, di fare coppia e famiglia; si consideri che l'ISTAT ha stimato che nel 2008 sono stati celebrati 246.000 matrimoni, circa 4 ogni mille abitanti. Per avere un'idea del radicale cambiamento - peggioramento, oserei dire - in atto nella società italiana basta ricordare che nel 1972 rispetto ai 246.000 di oggi, erano stati celebrati 420.000 matrimoni; ed i figli messi al mondo erano di più, più, pur se anche allora avevamo un tasso basso. Come se ciò non bastasse, i giovani, il futuro della nostra società, hanno pagato e continuano a pagare il prezzo della crisi economica; infatti, sempre secondo dati diffusi dall'ISTAT, il ricorso alla cassa integrazione, che è stato il principale e positivo strumento di sostegno sociale della crisi, ha provocato parallelamente la riduzione dell'occupazione giovanile; nel 2009 i giovani occupati erano 300.000 in meno rispetto al 2008. In sostanza, l'occupazione precaria ha pagato lo scotto della crisi economica e nel 2010 i dati sono peggiorati. Sempre in tema di occupazione, il Documento in esame conferma come nello scorso anno la crisi abbia continuato ad influire negativamente sul mercato del lavoro; nel 2010 il tasso di disoccupazione si è collocato all'8,4 mostra un timido ottimismo e stima che nel 2011 l'occupazione tornerà a crescere dello 0,5 per cento. Peccato, però, che nei primi mesi del 2011 le già timide e poco consolanti previsioni della maggioranza siano state smentite nei fatti. Voglio, infatti, ricordare che secondo l'ISTAT, in Italia, a marzo 2011, per il terzo mese consecutivo, il tasso di disoccupazione su base annua si è attestato all'8,6 per cento, lo 0,2 in più rispetto al 2010, questo smentendo le previsioni del Ministro. Sono numeri allarmanti, soprattutto se si considera che l'ISTAT ha rilevato che la disoccupazione giovanile si attesta al 29,4 per cento, un dato che è stato definito un record storico dal 2004 ad oggi. Vuol dire che un giovane su tre non ha lavoro e non ha la possibilità Che futuro ha questa società? Con questi dati alla mano, mi sento di affermare che il Governo ha inspiegabilmente sottovalutato il problema della disoccupazione giovanile, perché gli obiettivi delineati in questo Documento non sono capaci di contrastare questo triste fenomeno. Ci saremmo aspettati un vero e proprio «piano industriale», un progetto di riforma del lavoro e di rilancio dell'occupazione soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ma voglio essere ottimista voglio augurarmi che il Governo si ravveda su questo aspetto e affronti in modo serio e risolutivo le problematiche sopratutto legate al mondo giovanile. La disoccupazione dilagante, purtroppo, è solo un aspetto della grave crisi economica che ormai da tempo attanaglia il nostro Paese. Secondo il rapporto ISTAT sulla povertà in Italia, nell'anno 2009, erano 7.810.000 gli italiani che versavano in condizioni di indigenza e di povertà, con un reddito bassissimo, inferiore ai 983 euro mensili. Ma quelli che ne avevano 983, ne avevano già tanti! Secondo studi accreditati, questi dati sono confermati per il 2010. Il sentire popolare ci dice anzi che sono peggiorati. Il Documento di economia e finanza dedica un'apposita parte al «Contrasto della povertà», individuando la *social card,* come una delle soluzioni; sembra essere l'unica. sembra essere l'unica. Noi nutriamo delle perplessità su questa soluzione perché propone una sorta di *welfare* caritatevole che si traduce nell'erogazione di somme irrisorie

sul fisco familiare proprio non si è detto nulla. Si è preferito tacere perché è come se non ci si accorgesse che esiste un altro buco nero all'interno della nostra società. Vorrei concludere con una frase di Eleanor

italiani, siamo chiamati a creare le condizioni affinché la società tutta, ma soprattutto i giovani possano sognare e soprattutto realizzare i propri sogni. *(Applausi

a me sembra che la lettura di questo documento ci consegni una notevole sorpresa. Il Governo crede pochissimo, per non dire che addirittura non crede affatto, al federalismo fiscale. Mi sembra una sorpresa perché è una parola d'ordine molto sbandierata di cui si parla a ogni piè sospinto. Ho fatto un conto, perché a volte i dati quantitativi servono a capire anche la sostanza dei problemi. Su 416 pagine

relativa al Patto di stabilità interno e dieci righe nel Programma nazionale di riforma. Sono tra l'altro righe abbastanza misere, in cui si dice che si passerà dalla spesa storica ai costi e ai fabbisogni standard

Ci siamo astenuti su alcuni decreti legislativi, come l'ultimo relativo al fisco regionale. Abbiamo votato contro altri, come sul fisco municipale. Abbiamo votato a favore di altri ancora, come quello concernente l'ordinamento di Roma Capitale. Tuttavia noi crediamo nel federalismo fiscale e abbiamo contribuito a definire la legge n. 42 del 2009 in cui ci riconosciamo pienamente. Ci dispiace che la maggioranza e il Governo, che quella legge avevano voluto insieme con noi, non siano altrettanto convinti della sua bontà.

ad utilizzare la leva formidabile ed epocale che il federalismo fiscale della nostra Costituzione, se correttamente inteso, mette a disposizione.

nel Documento, che si chiama Carta delle autonomie locali, al momento in discussione al Senato. Essa potrebbe consentire risparmi fortissimi e migliore efficienza nel funzionamento della pubblica amministrazione, superando ad esmpio il dualismo

Noi vediamo un appuntamento molto importante nel prossimo decreto legislativo, quello relativo agli interventi speciali e alle politiche di coesione per il Mezzogiorno. Al momento manca completamente il raccordo

e che consentirà una verifica in Commissione circa il modo con il quale si vuole effettivamente mettere mano a questa riforma importante, correggendo anche

quella che negli altri Paesi europei nostri *partner* è una risorsa fondamentale: le città e le comunità locali come veicolo di

che davvero richiederebbero una diversa considerazione dei territori, delle città e delle Regioni, se davvero questa maggioranza e questo Governo credessero al federalismo fiscale, mentre, sulla base di questo documento, dimostrano di non averlo assolutamente a cuore.

sul quale sono già intervenuto in altre occasioni. Nel Documento viene messo in evidenza che le entrate nel 2010 derivanti dal lotto, dalle lotterie e da altre attività da gioco sono state di 8.129 milioni di euro e si prevedono, solo per la categoria lotto e lotterie, maggiori risorse per 104 milioni di euro. Questa è l'entrata erariale. A fronte di essa vi è una raccolta da gioco pari ad oltre 60 miliardi di euro, cui si affianca una raccolta illecita parallela che fa stimare la raccolta da gioco annuale in 100 miliardi di euro. euro. Il Governo nella legge di stabilità aveva denunciato il grave rischio che corre il nostro Paese, primo al mondo nella diffusione delle offerte da gioco, con il gravissimo fenomeno della ludopatia.

Sono soldi che vengono presi dalle tasche degli italiani.

e gioca nella speranza di vincere. I monopoli di Stato, che peraltro abbiamo ascoltato

è una grandissima sciocchezza: la verità è che la vincita viene dal giocatore reinvestita nuovamente nel gioco, quindi, continua ad esserci questa erosione dell'economia del cittadino, in un settore che rappresenta per lo Stato una forma di introito erariale con dei costi sociali elevatissimi, perché dietro questo fenomeno c'è la disperazione della gente, ci sono appartamenti ipotecati, negozi chiusi, prestiti, c'è l'usura, la criminalità organizzata che controlla il settore. Il nostro sta diventando uno Stato biscazziere, nel senso che utilizza

Avevamo presentato, ed è stato approvato all'unanimità dalla Commissione antimafia, un documento in cui invitavamo il Governo a rendersi conto che al settore del gioco al settore del gioco si connettono altri fenomeni criminali di grande importanza quali l'usura (che ho citato poc'anzi), l'estorsione, in modo particolare, e il riciclaggio. Oltre al dramma sociale, c'è il *business* della criminalità organizzata. Noi speravamo di trovare in questo Documento un'inversione di tendenza, invece la tendenza è quella di aumentare l'offerta da gioco, ossia offrire ai malati ulteriori occasioni di gioco, perché lo Stato deve lucrare sugli introiti erariali. Ma su quei 100 miliardi sottratti dalle tasche degli "ammalati", lo Stato poi prende 8 miliardi. Vi rendete conto dell'assurdità di questa politica, che incrementa l'offerta del gioco per ricavare una somma che rappresenta meno di un decimo di ciò che viene tolto dalle tasche degli italiani? Noi speravamo di trovare un segnale, una riga, una parola che impegnasse il Governo a ritrovare un'etica, nell'interesse dei cittadini, ad

Noi speravamo in un messaggio diverso, che invece non c'è stato, mentre per noi questo aspetto etico, che ha dei risvolti criminali estremamente pesanti, caratterizza tutto il Documento di economia e finanza. Noi speriamo in uno Stato che recuperi l'etica che abbia a cuore l'interesse dei cittadini, e non soltanto quello di far tornare apparentemente i conti, applicando attraverso forme

alcun riferimento al macrobiettivo contenuto nel Piano sanitario nazionale 2011-2013, che indica appunto nella salute e nel benessere delle persone e delle comunità un elemento di sviluppo, di coesione sociale e di innovazione,

esso viene trattato solo in rapporto alla razionalizzazione della spesa e alla riduzione dei costi, senza alcuna attenzione a coordinare questa razionalizzazione e riorganizzazione della spesa con quella innovazione che renda più appropriata la spesa e migliore la cura nel nostro Paese. I tagli lineari che sono stati fatti ed il blocco delle assunzioni hanno aumentato il precariato fra il personale medico e infermieristico. Oltre a ciò, c'è l'invecchiamento della popolazione medica e alla sua femminilizzazione, che avrebbero richiesto anche una diversa organizzazione del lavoro.

questa situazione viene risolta nel modo che le è proprio, quello cioè di pensare ad uno sblocco dell'accesso all'università, che finora prevedeva il numero chiuso, che dovrebbe essere pagato dagli studenti e dalle aziende ospedaliere.

di tutto il resto della popolazione medica. È necessario che il Ministro della salute e il Ministro dell'università prendano degli accordi affinché ci sia un raccordo diverso tra università e policlinici, tra policlinici e ospedali del territorio, riavvii una rivisitazione dei rapporti organizzativi ed economici tra insegnamento ed assistenza. Quindi, è una sfida che richiede innovazione e anche capacità di una *governance* diversa: *governance* diversa che ci viene richiesta soprattutto nelle Regioni del Sud del Paese, che sono chiamate ad attuare i piani di rientro e che dovrebbero poterlo fare

ma anche in rapporto ai cambiamenti epidemiologici che ci sono stati e, quindi, all'aumento forte della cronicità. Di questo non si fa alcun cenno e non c'è alcuna attenzione a definire con concretezza, per le future sessioni di bilancio, le dimensioni e le procedure degli interventi in conto capitale, in particolare per favorire la riorganizzazione delle reti ad alta specializzazione e delle tecnologie, e anche per favorire l'accesso ai servizi di eccellenza e ai percorsi di cura integrati per la prevenzione nel sistema distrettuale ospedaliero, per garantire uguale accesso ai cittadini di tutte le Regioni. Vorrei soffermarmi anche sul fatto che non si dice nulla di un investimento assolutamente importante per costruire un monitoraggio della qualità dei percorsi di cura. Questo sistema di monitoraggio è essenziale se vogliamo stabilire un modello diverso di *governance* di un sistema che si vuole profondamente federale e che di fatto rimane ancora centralista. l'Europa e l'Organizzazione mondiale della sanità ci chiedono di promuovere la salute in tutte le politiche, perché la complessità degli interventi per la prevenzione e per la cura non può essere affrontata solo nei settori verticali, verticali, cioè solo nel sistema sanitario, e per far questo l'Europa ci concede anche dei fondi. Non capisco come non si possano promuovere progetti di politiche integrate per favorire la salute quando ci sono anche le risorse a disposizione e l'Europa, in un sistema che vuole essere di riforma e di innovazione, ci chiede di farlo. Questo va nell'interesse di tutti i nostri cittadini, e mi auguro

com'è noto, il Documento di economia e finanza costituisce lo strumento programmatico, previsto dalla legge n. 39 del 2011, che si sostituisce alla Decisione di finanza pubblica, che a sua volta sostituì il Documento di programmazione economico-finanziaria. La legge n. 39, all'articolo 2, prevede che il DEF sia presentato ogni anno al Parlamento per consentirne l'esame e la successiva trasmissione al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, affinché possa divenire parte

nelle sue recenti decisioni. In particolare, le priorità indicate dal Consiglio europeo dello scorso 24 marzo prevedono il varo di un piano pluriennale di risanamento, precisi obiettivi in merito al disavanzo, alle entrate e alla spesa, la strategia per raggiungerli e un calendario di attuazione, che abbia cura di accelerarne gli esiti, soprattutto nei Paesi che versano in situazioni più difficili. Per quanto riguarda i piani di riforma per la crescita e l'occupazione, secondo il Consiglio europeo, gli Stati membri dovranno attuare, in particolare, misure atte a rendere il lavoro più attraente; aiutare i disoccupati a reinserirsi nei settori produttivi; lottare contro la povertà e promuovere l'inclusione sociale; investire nell'istruzione e nella formazione; conciliare sicurezza e flessibilità; riformare i sistemi pensionistici; attirare capitali privati per finanziare la crescita; stimolare la ricerca e l'innovazione; offrire un accesso efficace alle energie, sia in termini di costi, sia in termini di efficienza. Lo stesso Consiglio europeo ha inoltre approvato il Patto euro plus, al fine di realizzare un più stretto coordinamento delle politiche economiche per la competitività e la convergenza. Si tratta di un impegno stringente, che deve far sì che i diversi Paesi che utilizzano la stessa moneta non abbiano politiche economiche disgiunte e non armonizzate. Per quanto ci riguarda, il DEF prevede una diminuzione, tra il 2013 ed il 2014, del debito pubblico e un Programma nazionale di riforma che tenga conto del suo impatto, facendo sì che la proposta in esame risulti positiva sugli effetti che derivano sui conti pubblici, sul saldo tra risparmi di spesa e maggiori costi sostenuti, sul miglioramento delle finanze pubbliche. Secondo la previsione del DEF 2011, le dieci priorità dell'analisi annuale della crescita sono quelle che riguardano il risanamento di bilancio, la correzione degli squilibri macroeconomici, la stabilità del settore finanziario, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la riforma dei sistemi pensionistici, una maggiore facilitazione nel rientro dei disoccupati nel mondo del lavoro, una maggiore sicurezza e flessibilità nel lavoro, lo sfruttamento del potenziale del mercato unico, una maggiore attrazione di capitali privati destinati a finanziare la crescita, il destinati a finanziare la crescita, il miglioramento del mercato energetico e di risparmio di energia. A questi dieci punti il DEF collega le misure prioritarie connesse con gli impegni derivanti dal Patto euro plus. Si tratta, in particolare, della riforma fiscale, con l'allargamento dell'imponibile e la riduzione delle aliquote; dello sviluppo perequativo del Meridione d'Italia, attraverso una regia nazionale e misure fiscali di vantaggio;

della formazione permanente; del turismo; dell'agricoltura, con interventi di natura irrigua; della giustizia, con l'accelerazione delle varie procedure; della pubblica amministrazione, attraverso interventi di trasparenza, efficienza e semplificazione. Diceva Anton Cechov che è più facile chiedere ai poveri che ai ricchi. Ebbene, credo che le misure individuate dal Governo nel DEF 2011 non solo non creino aggravi particolari per le fasce deboli, ma mirano a migliorare l'efficienza dello Stato, il dinamismo del mercato, le opportunità di lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e materiali, attraverso strumenti ben armonizzati e suscettibili di ulteriore implementazione, capace, a sua volta, di migliorare proprio la situazione di chi vive condizioni di disagio. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, l'Italia è un Paese duale. Come ha più volte sostenuto il ministro Tramonti, in Italia la media della crescita, dello sviluppo, del debito, dell'occupazione non presenta elementi di armonicità. Detti parametri, anzi, risultano sperequati. È proprio in considerazione di tale situazione, pertanto, che l'auspicio che formulo non può che essere rivolto alla implementazione ragionata delle misure rivolte al Sud.

senza alcun pregiudizio né di tipo campanilistico, né di tipo politico, culturale, o peggio subculturale, come purtroppo talvolta accade. Ritengo che un moderno meridionalismo debba partire dagli errori compiuti, dalla loro ammissione, per non ripeterli, ma ritengo pure sia necessario evitare che se ne compiano di nuovi, che sarebbero letali ed acuirebbero il dualismo cui facevo prima riferimento. Il Sud, inteso sia come luogo geografico, sia come luogo economico e sociale, ha bisogno di semplificazione, di sicurezza,

Il Sud ha bisogno poi di una burocrazia competente, una burocrazia senza dubbi e senza prezzi. Ha bisogno di risorse per le progettazioni e di velocità nella spesa; ha bisogno di opportunità per i propri talenti e deve offrire affidabilità, efficienza, trasparenza, ordine, capacità di contrasto verso la criminalità, verso la clientela, verso pericolose sacche di privilegio, ormai del tutto intollerabili ed inconciliabili con le condizioni del Paese. Ma il Sud ha bisogno anche di sconfiggere i pregiudizi di cui è portatore o, anzi, vittima. Lo Stato, in tal senso, deve offrire, a sua volta, affidabilità e coerenza. Pertanto, la giusta lotta all'assistenzialismo non deve riguardare soltanto i lavoratori socialmente utili, diffusi al Sud, ma anche la cassa integrazione falsa o le quote latte, diffuse al Nord; non soltanto la mancata emissione di qualche scontrino, come accade al Sud, ma anche la falsa fatturazione o le false transazioni con Paesi incontrollabili, come accade al Nord; non soltanto la lotta al crimine manuale, ma anche a quello finanziario e a quello imprenditoriale, diffuso in tutto il Paese. Non credo sia necessario precisare meglio il senso di queste parole, anche perché non credo alla sterile polemica campanilistica. Credo, invece, che esse debbano diventare patrimonio comune dell'azione del Governo, così come patrimonio comune diventare il concetto, non solo enunciato, ma anche praticato, della perequazione infrastrutturale, indispensabile per raggiungere qualsiasi risultato in termini di riequilibrio armonico delle condizioni del Paese. I tagli orizzontali hanno salvato la nostra economia ed il nostro bilancio. Adesso, però, bisogna pensare a forme più spinte di riduzione dei costi della pubblica amministrazione, in grado di recuperare le risorse necessarie ed assicurare l'auspicata politica perequativa. Penso ad interventi di esternalizzazione e penso anche alla sussidiarietà orizzontale di funzioni pubbliche. Il concetto liberale di Stato non può essere uno slogan, ma di questo avremo modo di parlare in altre occasioni, che mi auguro giungano presto all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche. Questo DEF, e concludo, costituisce una delle mosse della partita. Adesso, però, la partita deve essere giocata fino in fondo, e soprattutto, deve essere vinta con la consapevolezza e l'impegno di tutti, magari abbandonando logiche di piazza piazza o da salotto, del tutto inconciliabili con l'emergenza che vivono il Paese e i nostri cittadini. Chi pensa che esistono problemi di altri che costituiscono opportunità per qualcuno un nemico del Paese, è un nemico della democrazia e va sconfitto con responsabilità e con decisione. Con le misure previste nel DEF e con le politiche di crescita che esso prevede, si compie il primo passo.

Per la crescita occorrono riforme strutturali e scelte di priorità per la destinazione delle risorse; occorrono azioni amministrative coerenti con gli obiettivi, concrete e autorevoli. Il Governo non è in grado di fare nulla di tutto ciò. Questo è il dramma del nostro Paese dove ci sono potenzialità molto grandi, intelligenze, cultura, creatività, un patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale straordinario.

e ad usarli come strumento per un consenso, tra l'altro assai calante, e come clava contro tutti coloro che hanno una visione diversa della politica e del Governo. Non sono condivisibili, ma sono inadeguate e sbagliate le indicazioni su istruzione e università contenute nei documenti in oggetto. Il sapere è, secondo la Strategia Europea 2020, la leva essenziale per una crescita inclusiva e sostenibile, una crescita con più coesione;

questo parametro, crolla al quint'ultimo posto, seguita solo da Estonia, Regno Unito, Portogallo e Polonia. E per il contrasto alla disuguaglianza, accanto alle politiche fiscali, occorrono politiche per il lavoro e, soprattutto, un investimento sul capitale umano. È questa l'indicazione europea ed è questo l'esatto contrario di quello che sta facendo l'Italia, così come dimostra il DEF 2011. L'Italia parte già da una posizione molto più svantaggiata rispetto agli altri Paesi europei per quanto riguarda la percentuale di PIL investita sul sapere.

hanno evidenziato la produttività altissima degli investimenti in istruzione. E tutti gli altri Paesi a maggiore sviluppo in Europa (Germania, Francia e Gran Bretagna), pur a fronte di piani di risanamento dei bilanci e a strategie di contenimento, hanno comunque incrementato le risorse destinate al sapere.

nulla per il precariato e per la prima infanzia, e nulla, infine, per l'aumento del numero dei laureati, sul federalismo scolastico e sul diritto allo studio. Lo so, ne sono consapevole, il nostro debito pubblico è elevato, ma la scuola e l'università hanno già fatto moltissimo in termini riduzione degli investimenti in questi settori. Concludo con un'interessante osservazione che ho trovato nell'intervento che il presidente Obama ha pronunciato quest'anno sullo stato dell'Unione. Parlando del debito pubblico degli Stati Uniti d'America e della necessità di contenere la spesa, ha affermato più o gli Stati Uniti sono come un aereo appesantito dai debiti e dell'eccesso di spesa, ma tagliare sull'istruzione sarebbe come iniziare ad alleggerire l'aereo gettando giù i motori. Ecco, è proprio quello che è stato fatto dall'Italia in questi anni ed è quello che l'Italia continuerà a fare, secondo le indicazioni di questi documenti, documenti, nel prossimo futuro. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Documento oggi all'esame dell'Aula rappresenta il documento di programmazione finanziaria, e di bilancio previsto dalla legge n. 39 del 2011 nell'ambito delle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il Documento di economia e finanza diviene così il principale strumento della programmazione economico-finanziaria che si articoli in tre sezioni: la prima espone lo schema del Programma di stabilità del nostro Paese, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. l'analisi e le tendenze della finanza pubblica e contiene i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali. La terza riguarda, invece, il Programma nazionale di riforma,

produttività, occupazione e sostenibilità delineati nella nuova Strategia Europea 2020. La prima sezione del Documento di economia e finanza evidenzia l'andamento dell'economia mondiale, che a fine 2010 registrato un rallentamento mentre per il 2011 si prevede una crescita economica globale del 4 per cento ed un'espansione del commercio mondiale pari al 7,1 per cento. Il Documento in esame prevede

per cento. Il Governo rivede in questo modo al ribasso le valutazioni del DEF, Documento di finanza pubblica, approvato solo a settembre 2010, dove il PIL per il 2011 era stimato l'1,3 per cento. Inoltre, come sappiamo, siamo abbondantemente sotto la media comunitaria. Basta citare la Germania che nel periodo succitato

e del 119,4 per cento nel 2013. L'indebitamento netto, che solo nel Documento di settembre era stimato cento, nel DEF è stimato a 2,7 per cento. Nel sistema produttivo questi dati si traducono in un pesante impatto occupazionale e purtroppo dobbiamo continuare a registrare l'assenza di politiche volte al rilancio del Paese. Non possiamo prescindere dal predisporre riforme strutturali che incidano, nel medio e lungo periodo, sia sulla componente qualitativa sia su quella quantitativa del prelievo fiscale e della spesa pubblica. Il Programma nazionale di riforma, contenuto nella terza sezione del Documento in esame, disegna solo in parte riforme future, piuttosto ripropone azioni già intraprese. È un elenco di misure generiche, senza indicazione delle specifiche misure indispensabili per rimettere in moto un Paese bloccato. Servono urgentemente misure strategiche per il settore primario. L'agricoltura italiana dimostra ormai da anni di essere attraversata da uno stato di forte crisi. I produttori registrano problemi sempre più acuti in termini di competitività e di reddito: si evidenzia un calo di produttività che investe direttamente comparti strategici, forti problemi anche in riferimento alla commercializzazione della produzione. Parole importanti vorrei spendere anche per il turismo italiano. Economisti, media, Parlamento discutono di crisi ma mai abbastanza di crisi del turismo, anche se questo settore contribuisce per oltre il 10 per cento alla formazione del PIL. Il Governo ignora la crisi del turismo e ha penalizzato la già scarsa competitività delle imprese ricettive istituendo la tassa di soggiorno. Secondo Federalberghi, il fatturato turistico delle vacanze di Pasqua nel 2011 è stato inferiore del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010. L'obiettivo di raddoppio del PIL del turismo, più volte indicato da questo Governo come obiettivo da raggiungere entro la fine della legislatura, sarà quindi difficilmente realizzabile. Non esiste un piano strategico: mentre i viaggiatori nel mondo sono cresciuti nel 2010 del 6,7 per cento, il flusso di visitatori verso l'Italia non accenna a riprendere quota. Sarebbe auspicabile che il Governo adottasse un piano strategico concreto, così da trasformare realmente il turismo italiano da opportunità a risorsa. Riguardo alle politiche energetiche

che ha dato risultati fortemente positivi, sia in termini ambientali che economici, il Governo ha dimostrato recentemente di non riconoscere l'importanza di questo settore

100.000 posti di lavoro. Auspico che le dichiarazioni del Governo di porre particolare attenzione all'incentivazione dell'utilizzo di energia rinnovabile nell'annunciato piano casa si

per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla compatibilità sostenibile. Al riguardo, cito pacchetti anticrisi, approvati anche dalla nostra Provincia, che contengono misure per il rilancio economico, la tutela dei posti di lavoro e i contributi per l'innovazione,

Mi preme evidenziare che solo un vero progetto orientato alla crescita, che comprenda anche un progetto sulla fiscalità di vantaggio, la detassazione degli utili reinvestiti, un serio intervento sulle liberalizzazioni, politiche sociali centrate sulla riduzione fiscale per le famiglie e un moderno sistema di ammortizzatori sociali, è in grado di rispondere alle difficoltà economiche e finanziarie che coinvolgono,